*(PD-Ulivo)*. Signor Presidente, dato il rilievo della materia, credo sia opportuno verificare, prima di iniziare la discussione, la presenza dei senatori nel numero richiesto per la validità della seduta.

verbale è approvato.

parte della circoscrizione che rappresento - persero la vita probabilmente anche più di 1.000 uomini e bambini, a causa di un'esplosione nelle viscere della miniera di carbone dove lavoravano. Di questi, 171 erano emigrati italiani, in particolare molisani, calabresi, abruzzesi e campani. Ma c'erano anche polacchi, irlandesi, russi e slovacchi. Gente povera e disperata, costretta ad emigrare dal proprio Paese nella speranza di trovare qualcosa di meglio per sé e per la propria famiglia. Ringrazio il Governo italiano, spronato e sostenuto in questo dal vice ministro e collega Franco Danieli, per aver contribuito con una donazione al restauro delle lapidi del cimitero in cui sono sepolte le vittime. Oggi avrei voluto essere anch'io con le centinaia di persone che si sono recate in pellegrinaggio a Monongah per commemorare il centenario e ricordare questi eroi, ma il dovere mi impone di essere qui per adempiere alle responsabilità del mio lavoro di senatore di quella circoscrizione. Signor Presidente, colleghi, desidero chiedere all'Assemblea di unirci anche noi a coloro che sono sul posto con un minuto di raccoglimento e di silenzio in memoria delle vittime di quella tragedia e di tutte le tragedie sul lavoro, dove essere umani di qualunque nazionalità hanno perso la loro vita. Credo di interpretare il pensiero di tutta l'Assemblea nell'associarmi alle parole del senatore Turano.

di Torino. Nello stabilimento della ThyssenKrupp, in Corso Regina, quartiere nuovo dove permane la presenza di un polo produttivo, vi è stato un grave incidente sul lavoro: l'esplosione - pare, al momento - di una camera all'idrogeno, utilizzata per la lavorazione dell'acciaio.

in Italia ha deboli disegni di investimento e di sviluppo e non investe più sulla sicurezza, sul mantenimento di buone condizioni di lavoro e di produzione.

fatto accaduto a Torino: ancora degli operai muoiono mentre lavorano. È la prima notizia che ci è giunta questa mattina. La domanda

Esiste una ragione? L'incuria, l'inosservanza delle norme o la scarsità dei controlli possono aver concorso a determinare questo come altri episodi tragici? Le chiedo, signor Presidente, che il Ministro del lavoro venga in Aula a riferire su questo episodio e ad indicare quali siano gli obiettivi, le scadenze e i programmi del Governo che puntino proprio proprio ad impedire le cosiddette morti bianche, che altri lavoratori sacrifichino la propria vita durante la prestazione delle loro difficili mansioni.

veramente inusitato. Sappiamo benissimo qual è il gioco di questa Aula, che credo sia delle aule parlamentari di tutte le democrazie del mondo. La maggioranza cerca di portare avanti il più rapidamente possibile i disegni di legge che ritiene opportuni

è di moda parlare anglosassone. In questa sede invece che cosa è accaduto? È accaduto che non c'è stato il solito autostruzionismo in qualche modo nascosto, che alcune volte viene avanti attraverso le dichiarazioni di parlamentari della maggioranza.

e la Nazione ci sente attraverso le radio, ci guarda attraverso le televisioni e ci legge attraverso i resoconti stenografici, credo che il presidente Finocchiaro debba dire

*(Aut)*. Mi associo, naturalmente, al ricordo del dramma. Da Torino stanno arrivando le seguenti notizie: un operaio è morto, altri nove sono rimasti feriti, e alcuni di essi sono in condizioni disperate.

c'è stata una fuga di olio combustibile. La squadra che operava di notte ha cercato in prima persona di spegnere le fiamme con gli estintori e con le manichette dell'acqua. L'esito è stato drammatico, perché ci sarebbe stata una reazione dell'idrogeno liquido a contatto con l'olio refrigerante. È il secondo, gravissimo, incidente;

la pressione sugli orari e la flessibilità hanno messo a rischio molte volte la salute dei lavoratori. È stato un dramma: la squadra è stata investita dall'olio bollente e l'esito è drammatico.

infatti, delle morti sui luoghi di lavoro, ma dobbiamo ricordare anche le morti di coloro che vengono ricoverati in ospedale e hanno bisogno di assistenza. Ciò avviene ogni giorno, dagli ospedali di Brescia a quello di Vibo Valentia, dove una ragazza, ricoverata

un mese fa tutta Italia è stata riempita di manifesti del Ministero della salute per il trentennale della legge n. 833 del 1978: un manifesto ridicolo, che parlava di amore e di perfezione tecnica.

vorrei che lei dal suo alto scranno richiamasse alla sua responsabilità il Ministro della salute, sempre disattento ai gravi problemi degli ospedali.

La classe politica deve reagire: non si può reagire soltanto quando c'è lo straniero, bisogna farlo quando la morte viene da noi, dal modo di lavorare. A mio avviso, il Senato, che ha dato storicamente prova di unità e compattezza in questa materia (dai tempi della Commissione Lama, fino al lavoro meritoriamente svolto dalla Commissione presieduta dal senatore Tofani) con l'approvazione di una normativa che, evidentemente, non è sufficiente, deve dare un segnale. Signor Presidente, chiediamo che il Ministro del lavoro venga urgentemente a riferire in Senato su quanto è accaduto e su cosa il Governo intende fare per porre fine alla vergogna delle morti bianche. Ci associamo, inoltre, alla richiesta che il Senato sia presente lunedì a Torino, sulla base della tradizione, che prima ricordavo, di attenzione a questo tema. La classe politica deve comprendere quello che accade nel Paese, la gravità di questo fenomeni, le ripercussioni che comportano. Oggi per 1.000 euro al mese si rischia di morire in fabbrica, signor Presidente, e so di parlare ad un interlocutore attento e che conosce questa tematica. Tutto ciò deve cessare. Per questo, signor Presidente, la preghiamo di dare seguito alle nostre richieste: il Senato sia presente a Torino e il Ministro del lavoro venga rapidamente a riferire in quest'Aula del Parlamento.

sono sicuro però che il Governo dovrà convenire sull'inaccettabilità di quanto sta accadendo. Signor Presidente, siamo abituati ormai, purtroppo, a discutere solo di leggi elettorali, di riforme costituzionali e di questioni molto lontane dai cittadini. La vicenda calabrese è qualcosa che fa rabbrividire. Vi mostro una pagina dei giornali di oggi, ma potrei mostrarle tutte, su cui compare

ma questo è inaccettabile. Mi è capitato, ministro Turco, precedendola nel suo alto incarico, di essere investito dall'onda di critiche riguardanti gli ospedali siciliani

leggo da «La Stampa», il giornale della sua città: «Lo scandalo di Vibo Valentia: una lunga storia di malaffare e di malavita». L'incredibile è che tutti sanno e nulla accade. Anzi, si alza il vice presidente della Giunta regionale, Vincenzo Spaziante, e si arrabbia pure, dicendo di non accettare che si parli di malasanità in Calabria. Ministro, chiuda la bocca a questo assessore irresponsabile. Presidente, il Gruppo dell'UDC desidera esprimere la più profonda solidarietà per il dramma accaduto stanotte a Torino. Ciò che ha detto la collega Alfonzi è l'esatta espressione di un sentimento che condividiamo. Riteniamo che il problema delle morti cosiddette bianche non possa dividere il Parlamento della Repubblica.

emettere provvedimenti di prevenzione nei confronti delle cosiddette morti bianche. Non sappiamo se il Governo ha fatto nulla; onestamente, in quel provvedimento non erano previsti neanche i fondi necessari per la prevenzione.

per il bene politico del nostro Paese. Il Gruppo dell'UDC esprime solidarietà specifica nei confronti delle persone drammaticamente ferite e ovviamente solidarietà ai familiari delle persone morte. La morte sul posto di lavoro è una tragedia enorme che ci riguarda direttamente, signor Presidente. *(Applausi dei

già citato da altri colleghi, credo che il Senato avrebbe non solo il diritto ma il dovere di inviare la Commissione competente a compiere visita

*interna corporis*, ma, in casi come questo, per poter aprire veramente un'indagine ed un'inchiesta serrata con una visita immediata sul posto.

relativo al Testo unico sulla sicurezza e a che punto sono gli impegni assunti dal Governo per il potenziamento dei servizi ispettivi. Per quanto sollecitato dal senatore Martinat, noi decideremo (non ho dubbi che in questo senso il Presidente della Commissione infortuni e morti bianche sarà concorde), di fare un'indagine specifica anche come Commissione e in tempi brevi. Il problema, però, Presidente e colleghi, è che gli infortuni, in alcuni casi e in particolare questo infortunio, avvengono in un settore, quello delle acciaierie, che ne è particolarmente soggetto. Abbiamo già fatto una verifica all'ILVA di Taranto, ma dopo la privatizzazione della Texid e la vendita ai privati delle acciaierie, gli infortuni sono enormemente aumentati. In più, in questo caso, vi è il sospetto che avendo deciso la ThyssenKrupp di chiudere lo stabilimento

Presidente, oltre a esprimere solidarietà, in generale rispetto ai morti sul lavoro, lei proponesse un minuto di silenzio e di raccoglimento in ricordo delle vittime, che continuano ad essere tre o quattro tutti i giorni. *(Applausi

anche in questa circostanza farà il proprio lavoro con impegno, approfonditamente, per capire cosa sia accaduto e quindi per proporre al Parlamento e al Governo iniziative per

«siamo rammaricati, siamo distrutti dal dolore»; diciamo anche che ci sono meccanismi perversi che stanno creando limiti ad azioni di prevenzione, di conoscenza e di informazione.

vista la gravità di taluni feriti; dobbiamo pure chiaramente assumere una iniziativa di responsabilità, attribuendo poteri specifici

intervengo per esprimere, a nome mio e del Gruppo Sinistra Democratica, il cordoglio e la vicinanza ai familiari della giovane ragazza morta a Vibo Valentia in un evidentissimo caso di malasanità e per esprimere, al tempo stesso, una profonda indignazione. Questa mattina, già in Commissione sanità, ho posto il problema chiedendo che il Ministro della salute venisse a riferire in Commissione sull'esito delle

e per fare il punto su una situazione evidentemente intollerabile. Vorrei ricordare che quell'azienda sanitaria è stata investita da una inchiesta giudiziaria su infiltrazioni mafiose e che su quella

il Governo faccia un atto straordinario per intervenire e mettere ordine ad una situazione non più tollerabile.

di destra avrebbero pensato e sappiamo che, quando si preme troppo l'acceleratore sulla competitività, sulla produttività, eccetera, si rischia di perdere di vista l'altra parte della componente

L'episodio è particolarmente grave proprio perché si tratta di un'azienda che doveva essere trasferita e tutto fa supporre che qualcosa non sia più seguito con la necessaria attenzione. Mi associo quindi alle proposte di intervento del Ministro,

approvato una legge importante che deve trovare applicazione e tuttavia le morti continuano ovunque: credo debba essere richiamata l'attenzione sulla pressione enorme che c'è oggi sul mondo del lavoro. Le leggi vigenti, ovverosia le leggi non scritte ma dominanti del sistema produttivo, sonoflessibilità, disponibilità, straordinari, produttività accresciuta la pressione dal punto di vista delle condizioni del lavoro e degli orari di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori diventano via via più insopportabili. Di questo sistema produttivo si muore: dovremmo prendere

che, anche di fronte a situazioni che palesano questa criticità, questo cortocircuito istituzionale, il Parlamento avvii immediatamente un dibattito serio sulle riforme costituzionali al fine di pervenire ad una razionalizzazione

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale intervengo a proposito dei fatti di Vibo Valentia per ricordare che già nell'occasione del gravissimo caso accaduto all'inizio dell'anno la Commissione si recò in quella struttura e constatò una drammatica situazione, ma di fronte al problema di coscienza se chiudere quell'ospedale, come molti chiedevano, lasciando però privi di assistenza sanitaria oltre 200.000 cittadini, si scelse la strada di fare alcune prescrizioni molto importanti che, per la verità, sono state

che vede le morti durante i trasporti (oltre tre durante l'anno; ricordiamo il caso gravissimo del bambino deceduto poco tempo fa), che pone problemi di truffe gravissime, di omicidi.

associo alle condoglianze e al dolore espressi dai colleghi e dalle colleghe nei confronti delle famiglie colpite dalla morte stanotte a Torino. stata sollecitata la presenza del Ministro del lavoro e mi sembra giusto. Voglio dire però che in quanto Ministro della salute ho ritenuto di assumere il tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro come una priorità del mio Dicastero. Abbiamo lavorato d'intesa con il ministro Damiano e, pur in attesa della presenza del Ministro che fornirà elementi più dettagliati, posso dire che gli atti applicativi della legge delega per la tutela della salute nei luoghi di lavoro luoghi di lavoro sono in via di definizione, che nella legge finanziaria sono stati stanziati 50 milioni di euro proprio per rendere applicativi tali atti e che è entrato in vigore il patto siglato dal mio Ministero con le Regioni italiane per potenziare gli atti ispettivi delle ASL nei luoghi di lavoro. Ovviamente l'accaduto così grave ci sollecita a rendere ancora più stringenti le iniziative già concordate. Per quanto riguarda la morte della ragazza a Vibo Valentia, ho vissuto questa notizia come davvero agghiacciante. Posso dirvi che la seguo con tutta la passione umana, la passione di una madre, la stessa passione che ho portato nel seguire lo scorso anno la morte di Federica. Ho seguito passo a passo la vicenda di Vibo Valentia dopo la morte di Federica e, ironia della sorte, proprio oggi al Ministero della salute sigleremo l'accordo con la Regione Calabria

So bene, però, che questo non basta. Discuterò, come ho fatto nel caso di Federica, con i genitori e con le autorità locali su che cosa fare. Mi è stato detto di adottare

di quanto sia inaccettabile che nel nostro Paese, nel nostro sistema sanitario, nel giro di un anno si muoia per appendicite e per tonsille. Ripeto che ciò è inaccettabile! Quindi, con questo sdegno, con questa passione e con la tempestività e l'impegno che rivendico nel corso dell'ultimo anno e mezzo, continuerò il lavoro svolto.

grazie, senatore

Diversi Gruppi ieri hanno esaurito i tempi a loro disposizione per l'esame del decreto-legge al nostro ordine del giorno. Oltre a ciò, la Presidenza ha bene a mente che, ai sensi dell'articolo 78, comma 5, del Regolamento, essendo scaduti i trenta giorni per l'approvazione del decreto-legge,

Per evitare di ricorrere a tale mezzo estremo, e consentire ai Gruppi di potersi pronunciare sulle rilevanti norme al nostro esame, la Presidenza - come ha fatto altre volte - consentirà ai Gruppi che abbiano esaurito i loro tempi una dichiarazione di voto, per due minuti, su ciascuno dei testi che verranno posti in votazione. I senatori dei Gruppi che hanno esaurito i tempi che intendono esprimere il proprio dissenso rispetto alle posizioni del Gruppo di appartenenza o esprimersi per annuncio di voto

che si propone di estendere e rafforzare la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e, la libera circolazione e il libero soggiorno una delle libertà fondamentali da esercitare nell'Europa come spazio senza frontiere e per l'esercizio di una cittadinanza che la direttiva indica come *status* fondamentale, da riconoscere a chiunque è membro di uno degli Stati comunitari. La direttiva dice anche che va superato ogni carattere settoriale e frammentario delle norme tra gli Stati; figuriamoci - a proposito anche di quello che sta avvenendo nel nostro Paese - se possiamo consentirci norme

indica anche che si deve applicare un trattamento più favorevole non solo ai lavoratori, ma anche ai richiedenti lavoro, persino dopo i tre mesi, in rispondenza a precise disposizioni della Corte di giustizia europea.

presso i luoghi di residenza nel caso di richiesta di permessi di soggiorno prolungati o addirittura della residenza. Si dice, inoltre, che i documenti richiesti per questo adempimento devono essere indicati in modo tassativo e devono avere caratteri tali da evitare di prestarsi a interpretazioni e pratiche cosicché l'adempimento di questa formalità amministrativa possa diventare ostacolo all'esercizio della libera circolazione del soggiorno. Se queste sono le corrette interpretazioni degli articoli della direttiva europea in oggetto (cioè il 5, il 6 e il 7), l'emendamento qui proposto è chiaramente

Presidente, mi permetta

al senatore Garraffa, che si permette pure di fare una ramanzina, quasi che fosse lui il Presidente di questa Assemblea. A noi di ciò che scrivono i giornali sulle sconfitte dell'Unione non interessa assolutamente nulla. Questo deve essere chiaro.

dà a tutti la percezione che, essendo divisi pressoché a metà, per garanzia reciproca - perché può capitare da una parte e dall'altra - le votazioni debbono cercare di essere svolte ordinatamente.

Su questo argomento, però, abbiamo sperimentato qualche volta già il metodo di stare tutti

né ad affermazioni pesanti, non avendo peraltro il microfono a disposizione. Collega Garraffa, glielo dico pacatamente: la violenza verbale che lei utilizza fuori dagli interventi ufficiali, ma adesso anche nel suo intervento, ha voluto sottolineare un aspetto disdicevole per l'Assemblea. Lei ha voluto dire che ieri le cadute del Governo, che pure hanno avuto luogo, sono state causate da voti non esistenti. Questo è inaccettabile, senatore senatore Garraffa, per il Presidente; altro che ritirare o no una scheda. Ieri il Governo è andato sotto perché non avete i numeri e non riuscite a prenderne atto.

e, non essendo tra quelli che grida (ed è noto a tutti), dico pacatamente che è inaccettabile ciò che lei poco fa ha sostenuto. Invito la Presidenza - perché non posso rivolgermi a lei,

Cito le parole del Capo dello Stato, pronunziate ieri a Milano. Per affrontare i temi della sicurezza il Presidente della Repubblica consiglia di usare la chiave cooperativa e non conflittuale, perché quella della condivisione è la via più consigliabile e può risultare la più produttiva. È un messaggio che noi giriamo a voi, colleghi della maggioranza; noi lo abbiamo raccolto fin dall'inizio. Abbiamo tentato in tutti in modi di contribuire al miglioramento di questo testo, non facendo ostruzionismo. Avete sino ad oggi rigettato le nostre proposte migliorative e non conflittuali, soltanto perché una parte della vostra maggioranza è condizionata dalla sinistra, che pone l'intangibilità di questo testo per la sopravvivenza del Governo. Noi ci inchiniamo dinanzi a queste parole del Capo dello Stato, che sono parole di grande saggezza; voi purtroppo non le state rispettando e di questo ci dispiace molto. Mi auguro, signor Presidente,

Vorrei sapere perché questa mattina la maggioranza ha chiesto il numero legale. Non è stata data nessuna risposta. Adesso, invece, si vuole partire velocemente per votare. Si tratta di una questione politica sulla quale l'Aula credo

nessun timore a rispondere al presidente Castelli. Come è ovvio e come è accaduto migliaia di volte nella storia parlamentare di questo Paese, se la maggioranza ha bisogno di venti minuti per mettere a punto un accordo, fa mancare il numero legale, punto. *(Commenti dal I discorsi del presidente Schifani sono assolutamente condivisibili sotto il profilo del merito e sotto il profilo del richiamo all'autorevolissimo del Presidente della Repubblica. Peccato che il comportamento di questa opposizione per tutta la giornata di ieri, e ancora oggi, sia stato assolutamente incoerente con quella nobile proclamazione di princìpi.

del senatore Mantovano, come del senatore Nitto Palma e degli altri colleghi dell'opposizione, abbiano fornito un contributo di merito di grande spessore e significato. Certo, ci aspettavano dalla maggioranza la ricerca di questa condivisione. La verità è che la maggioranza, nonostante gli interventi urlati del senatore Garraffa, ricerca la condivisione, ma solo tra

Pertanto, se il centro-sinistra voleva ricercare la condivisione nei provvedimenti, avrebbe tentato in tutti i modi di raccogliere il senso dei nostri interventi e quello che avevamo sostenuto. Voglio concludere invitando all'attenzione, è a tutti evidente che la crisi numerica in quest'Aula è determinata dai comportamenti di alcuni componenti della maggioranza maggioranza che, a turno, diventano o un pericolo per la tenuta del Governo, o un mito. L'ultimo al quale assistiamo - e non voglio citare la decisione di voto di ieri della senatrice Thaler - è il collega Dini, che fino a qualche tempo fa era guardato come fumo negli occhi, mentre ora siamo arrivati al punto che viene citato anche come un'ottima figura di Presidente nel dirigere i lavori Questa è la realtà nella quale si trova la maggioranza che tenta in tutti i modi di non far esplodere contraddizioni, evidenti per l'Assemblea, che peseranno sul provvedimento, come stanno facendo e come stiamo registrando.

Un attimo solo,

Mi dispiace, perché chiunque abbia sostenuto questo ha detto il falso: infatti il sottoscritto, che partecipava ad una riunione, è rientrato in Aula, ha votato e numerosi colleghi mi hanno visto.

intervenire. Chiedo ai colleghi un attimo di attenzione. Secondo la direttiva europea, il soggiorno e la circolazione dei cittadini dell'Unione, nei primi tre mesi, è completamente libera. L'unica condizione che lo Stato ospitante può imporre è quella di una dichiarazione di presenza da effettuare entro un congruo periodo

affermare, come si afferma nell'emendamento 1.300, che dalla mancata dichiarazione di presenza, che deve essere effettuata evidentemente prima cioè in un periodo che si pone prima dello scadere dei tre mesi, consegua l'idea, la presunzione che il soggetto si trovi in Italia da oltre tre mesi, significa allegare ad una facoltà un effetto sanzionatorio, ma principalmente significa incidere direttamente sul dritto di circolazione libera nei primi tre mesi. A mio avviso è una violazione della direttiva. Dopo di che vorrei dire un'ultima cosa: sia chiaro per tutti che quand'anche dovesse passare l'emendamento 1.300, quando vi troverete davanti un cittadino dell'Unione che non ha fatto la dichiarazione (e dunque voi presumerete si trovi in Italia da oltre tre mesi), e che sicuramente non farà

Signor Presidente, volevo segnalare che nella fila dei senatori Azzollini e Pisanu ci sono sette schede, se si va a controllare hanno votato per sette. Chiederei che la scheda accanto al senatore Santini venga tolta per cortesia.

con urla e strepiti che si susseguono e che rendono assolutamente poco prestigiosa l'Aula della quale facciamo tutti quanti parte. Sono convinto, Presidente, e penso che lei potrà sicuramente convenire, che i nostri Segretari di Presidenza, tra l'altro tutti molto bravi e attenti, dispongano di risorse economiche aggiuntive, emolumenti aggiuntivi per svolgere il loro lavoro apprezzato, dispongano di auto di servizio,

colleghi, se il cittadino omette di dichiarare la propria presenza, si presume che sia presente da oltre tre mesi.

Vi è la possibilità di allontanarlo dall'Italia? Secondo la vostra legge assolutamente no. State quindi scrivendo dei princìpi da buttare in faccia demagogicamente alla cittadinanza, senza alcun costrutto. Perché la realtà di queste cose, per voi che siete sotto la pressione della sinistra radicale, è di favorire una falsa e strumentale demagogia solidaristica rispetto alla sicurezza dei cittadini italiani. *(AN)*. Signor Presidente, questo emendamento è la cifra interpretativa dell'intero decreto-legge, nel senso che è la sintesi dell'inutilità. Questo decreto‑legge non serve a nulla. Lo ha confermato il ministro Amato nel momento in cui ha parlato di 200 provvedimenti di allontanamento; ha però trascurato un dettaglio: precisare che di questi 200 provvedimenti solo 40 sono stati di allontanamento effettivo e questo emendamento recepisce, sì, il comma 5 della direttiva che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, aveva omesso di recepire, ma lo recepisce male, indicando una semplice facoltà e non un dovere, come invece prescrive la direttiva medesima. Poiché non credo che il Senato debba essere impegnato nell'approvare degli emendamenti e dei decreti truffa, virtuali, privi di qualsiasi consistenza e di qualsivoglia riscontro concreto, annuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale.

abbiamo a lungo discusso di questo punto, cercando di fare in modo che la ragione prevalesse su posizioni assolutamente pregiudiziali, e di spiegare ai colleghi della destra che hanno sottoposto alla nostra attenzione il tema dell'attestazione della residenza anagrafica, come si trattasse di un tema inutile ed improponibile. Inutile, perché mancando la data certa della presenza in Italia, nessuno avrebbe mai potuto accertare il decorso dei tre mesi, a seguito dei quali sarebbe scattato l'obbligo dell'attestazione della residenza anagrafica; improponibile, perché si faceva discendere da quella attestazione di residenza delle sanzioni, come addirittura l'espulsione, cosa espressamente vietata tanto dall'articolo 27 della direttiva, quanto dal numero 11 dei *consideranda*. Tutto ciò premesso, abbiamo detto ‑ e il Ministro dell'interno lo ha spiegato a chiara voce in quest'Aula ‑ che il tema della data certa dell'ingresso dei comunitari in Italia può essere risolto solo con la modifica della direttiva. In questo senso lo stesso Ministro dell'interno ha chiesto in quest'Aula di avere un mandato chiaro in questa direzione e in qualche modo la conversione del decreto conferirà quel mandato che il Ministro dell'interno ha chiesto. Ci siamo industriati per cercare una soluzione che nell'ambito della direttiva e del trattato consentisse egualmente di poter addivenire ad alcune conclusioni che si ritenevano importanti. La prima soluzione che abbiamo trovato è stata quella di dire che, premesso che rendere generalizzato l'obbligo - così come si proponeva - prevedendo che tutti i comunitari avrebbero dovuto dichiararsi nel nostro Paese, avrebbe significato introdurre un principio per cui 30 o 40 milioni di turisti comunitari avrebbero fatto le file dinanzi ai nostri commissariati, una cosa che non aveva nessun senso logico oltre che una totale impraticabilità, con un grave danno per la nostra economia turistica. Abbiamo così individuato un meccanismo che rende facoltativa la dichiarazione di presenza, ma allo stesso tempo ne fa discendere delle conseguenze giuridiche, quali l'inversione dell'onere della prova, una presunzione *iuris tantum*, superabile della prova contraria, che questo cittadino comunitario stia in Italia da oltre tre mesi.

sull'ammissibilità - che la collega Thaler Ausserhofer molto opportunamente, richiamandosi proprio all'emendamento 1.300, ha detto che può essere assolta anche attraverso la dichiarazione di presenza all'interno delle strutture alberghiere, una misura che evidentemente aiuta gli organismi di polizia, aiuta il nostro Paese a dare quella prova della presenza, ad escludere coloro che sono in Italia per turismo dal novero dei controlli che invece dobbiamo svolgere per chi sta in Italia o intende stare in Italia più di tre mesi. Signor Presidente, questa è la soluzione massima, questa è la soluzione migliore che possiamo adottare nel rispetto della libertà di circolazione e di soggiorno prevista dal trattato, quindi assolutamente inderogabile, e nell'ambito dei principi della direttiva n. 38 del 2004, che non possiamo in alcun modo violare perché la nostra Costituzione non ce lo consente. E' evidente che, se cercheremo in futuro di modificare quella direttiva, potremo introdurre quel principio della data certa che ci consentirà di dare più chiarezza alla materia. È però del tutto evidente, signor Presidente, che

diritti, ma voluta dall'Unione europea proprio per garantire quei diritti di libertà e di soggiorno che noi in questo momento stiamo cercando di limitare in qualche misura ed è per questo che nascono le contraddizioni. Credo tuttavia che con un po' di buona volontà in quest'Aula e soprattutto nel rispetto dei suddetti princìpi,

Pensiamo che la sicurezza debba coniugarsi e contemperarsi con libertà e giustizia, che debba essere sicurezza nel diritto e sicurezza dei diritti, di tutti: di tutti: dei cittadini italiani, di quelli comunitari, degli esseri umani, uomini e donne, perché nel diritto internazionale i diritti fondamentali, tra cui quelli della libertà

poco fa: questa direttiva e il decreto che la attua per il nostro Paese ha come prima finalità quella di rendere la circolazione nel territorio europeo libera, non limitata e non vincolata,

*(LNP)*. Signor Presidente, con le disposizioni del Parlamento europeo non si dice alle Nazioni di rinunciare alla propria sovranità. Con l'emendamento 1.300, assolutamente risibile, che non garantisce nulla, è evidente la rinuncia alla sovranità su tutto ciò che riguarda l'ingresso clandestino di cittadini sia comunitari che extracomunitari.

poiché noi del Gruppo della Lega siamo stati eletti a rappresentare soprattutto i cittadini del Nord, insieme poi a tutti i cittadini italiani, ci chiediamo se in quest'Aula vi sia qualcuno che fa riferimento a potenziali elettori che arrivano da altre parti d'Europa e da altre latitudini.

voi non siate più in grado di gestire l'Assemblea del Senato, e che siate arrivati al punto di rinunciare in modo sfacciato alla vostra sovranità, non soltanto a livello

procediamo secondo criteri di snellezza perché abbiamo tempi stretti; per altro verso, l'interventismo

noi parlamentari non saremmo stati ostaggio di quest'Aula, come lo siamo stati, ma sarebbe stato ostaggio di una parte di questo ramo del Parlamento l'intero Senato, vale a dire l'istituzione camerale più alta delle nostre istituzioni democratiche. Siamo stati presi in giro da un gruppo che sapeva

nessuno Ci stiamo prendendo in giro! È una concessione alla posizione libertaria e lassista di Rifondazione Comunista e gli effetti sul nostro Paese, quando si verificheranno nuovi reati come quelli avvenuti nella città di Roma, saranno veramente devastanti.

all'ipocrisia. All'indomani del delitto della signora Reggiani furono sparse tante lacrime da parte del mondo politico. Il *Premier* della Romania ebbe la faccia tosta di dire che nel suo Paese la criminalità era diminuita

che di qui a qualche minuto annuncerà la richiesta di un ignobile voto di fiducia - che il suo Governo porta tutta intera la responsabilità del sangue che continuerà a scorrere nel nostro Paese.

ci sono state le dichiarazioni di voto e abbiamo votato i subemendamenti; mi auguro che non si abbia il cattivo gusto di non lasciarci votare neanche l'unico emendamento in campo in questo momento. momento. Mi auguro che la richiesta della fiducia, quando verrà, sia successiva all'unico voto che dovremmo fare. Avrei auspicato, da parte sua, il ricorso a strumenti come la ghigliottina, piuttosto che togliere, dopo che è stata

Signor Presidente, a nome del Governo, espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi

voluto trovare un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. Non è stato possibile: si è visto concretamente, anche ieri, nello svolgersi dei lavori d'Aula e, prima, nell'impossibilità stessa da parte della Commissione di concludere e nominare un relatore. A questo punto, il Governo ritiene debba essere assicurata la coerenza complessiva del provvedimento che ha concordato con la sua maggioranza. Il decreto, inoltre, deve essere ancora esaminato dalla Camera, dove è in corso la sessione di bilancio. Per questi motivi, abbiamo il dovere - e intendiamo esercitarlo - di assumerci la responsabilità di Governo in un tema tanto delicato.

prendiamo atto del definitivo fallimento della politica di questo Governo anche su un tema come quello della sicurezza.

questa fiducia viene posta contro i colleghi della stessa maggioranza. L'articolo 78 del nostro Regolamento, al comma 5, prevede la possibilità, per la Presidenza ed il Governo, di invocare questa norma, in forza della quale, nella giornata di oggi, si sarebbe potuto mettere in votazione

la fiducia al Governo

vorrei rivendicare la possibilità di esprimere un'opinione sulla fiducia e una convinzione diversa per quanto riguarda il merito del provvedimento. Si tratta di una palese violazione del nostro Regolamento che nemmeno la Conferenza dei Capigruppo può sanare.

Le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono state già comunicate ai Gruppi. Do ora la parola al Presidente della 5a Commissione permanente, senatore Morando, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.1000. Signor Presidente, nella riunione della Commissione, che si è

che avevamo singolarmente esaminato sia per la formulazione del parere della Commissione, sia in altri casi per la formulazione del parere sugli emendamenti all'Aula. Si tratta di emendamenti, signor Presidente, sui quali, ad uno per uno, avevamo espresso parere di nulla osta. Naturalmente, il nostro parere non può essere diverso adesso che quegli emendamenti li abbiamo esaminati non più ad uno per uno, ma tutti assieme, come componenti dell'emendamento complessivo del Governo, presentato per apporvi la questione di fiducia. Quindi, complessivamente il nostro parere sull'emendamento 1.1000 è di nulla osta, in coerenza con il pronunciamento della Commissione sui singoli emendamenti in sede di esame degli stessi per l'Aula.

intervenendo per primo nella discussione generale, all'inizio, avevo auspicato che, nel corso dei lavori, il decreto-legge sulle espulsioni fosse reso quanto più possibile conforme innanzi tutto al dettato costituzionale, poi alla direttiva comunitaria ed infine anche allo spirito comunitario che considera la libertà, la giustizia e la sicurezza pilastri dell'Unione Europea. Avevo auspicato che i temi della sicurezza, della giustizia e della libertà fossero coniugati, non essendoci un ordine di priorità,

alcuni tratti di discrezionalità che rendevano incerti e vaghi i comportamenti ai quali dovevano conformarsi i cittadini comunitari

stata abbandonata qualsiasi idea di legare la sorte dei comunitari a pregressi comportamenti o a misure

accettato, anche con una certa estensione - che tali provvedimenti fossero sottoposti ad un sistema di controllo giurisdizionale, affidato non più ai giudici di pace,

sottoposti ad una verifica discrezionale del potere esecutivo. I due problemi si legano perché, ottenuta una certa tassatività,

lo abbiamo ottenuto perché non c'è un riferimento specifico e obbligatorio alla detenzione nel CPT: una detenzione amministrativa odiosa che noi combattiamo da anni e che speriamo poter non dico eliminare del tutto, ma ridurre al minimo con i prossimi provvedimenti legislativi. Ciò è importante perché si tratta oltre che della vita di soggetti extracomunitari anche della vita di

delle possibilità di riduzione della detenzione nei CPT perché si dice che il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea. Che vuol dire ciò?

esasperati perché il numero di questi cittadini è abbastanza ridotto. Questa formula, secondo noi, apre una possibilità di trattativa della difesa, delle associazioni, di coloro che si interessano a questi cittadini per poter anche ottenere che il trattenimento non sia, per esempio, disposto per un CPT, che magari è lontano 100 chilometri dal luogo in cui

ci sarebbe piaciuto - ormai la polemica è alle nostre spalle - che questo provvedimento non venisse estrapolato dal pacchetto sicurezza e venisse mantenuto come disegno di legge. Ciò avrebbe consentito innanzitutto una più serena discussione in questa Aula e poi avrebbe consentito una discussione, una preparazione ed un'elaborazione molto più pacata, ragionata e meno traumatica in Commissione, ovviamente a fasi invertite: prima in Commissione e poi in Aula. Sarebbe stato, però, di grande aiuto per tutti (per il Governo, per l'opposizione e per la maggioranza). Ormai, siamo qui, di fronte a questo decreto, emendato e sottoposto a fiducia:

non vi sia più quel pericolo di espulsione di massa e che i lati odiosi di questo provvedimento, così caduti, non facciano gridare, all'esterno, ad un

che sono delle persone, non dei cittadini (come dirò poi meglio più avanti). Diritti universali e inviolabili della persona umana, come recita la nostra Costituzione.

non sia una preoccupazione nostra, della sinistra e, in modo specifico, della forza politica di cui faccio parte: lo è senz'altro,

Vi sono modi efficaci di rispondere sul tema della sicurezza, anche conformi, però, alla nostra storia, alla nostra identità di popolo e Paese democratico, al nostro diritto. Questo decreto - sul quale ci pronunciamo oggi - era segnato da qualche peccato originale. non ci interessa entrare nella polemica stucchevole se sia stato scritto su richiesta o sotto dettatura; questo Senato ne ha riconosciuto - secondo le

quanto alla conformità alla normativa europea ed alla nostra stessa Costituzione. Abbiamo esposto nel dibattito le nostre ragioni ed i nostri argomenti:

una nozione che si va costruendo ed affermando, anche con fatica. È questo un terreno che costituisce uno dei veri fondamenti dell'esperienza europea che oggi viviamo. La libera circolazione delle persone è certamente uno dei mattoni fondamentali dell'edificio che stiamo cercando di costruire.

Quando nella direttiva si dice che non si possono prendere provvedimenti limitativi in termini generali e generici ma che bisogna guardare ai comportamenti specifici

giuridica vede su binari paralleli l'uomo e il cittadino. Dalla rivoluzione francese in poi noi vediamo queste due diverse figure:

Da più di due secoli, dalla rivoluzione francese in poi, vediamo che esiste un patrimonio di diritti di tutele giuridiche, di protezioni che fanno capo ad un tempo all'una e all'altra figura. Questa è una concezione che si è tradotta direttamente nella nostra Costituzione, in particolare all'articolo 2 dove il concetto dei diritti inviolabili esprime esattamente questo principio, ossia che le tutele riguardino la persona umana in quanto tale e non certo per la sua appartenenza ad una realtà statuale.

conformità, alla Costituzione ed alla direttiva europea, più solida e più sicura. Non è il decreto che avremmo scritto noi! Probabilmente,

guardando alla repressione, ma piuttosto all'efficacia della presenza delle forze dell'ordine. Quindi, investendo risorse consistenti sulla sicurezza, dando risposta finalmente - cosa che non siamo mai riusciti a fare in questo Paese - alla domanda di coordinamento di forze all'ordine che forse quantitativamente sono anche in numero adeguato ma che certamente, per gelosie

aggiungere risposte diverse, perché non basta garantire la sicurezza quando ci sono milioni di famiglie che scivolano sotto la soglia della povertà, e tanti che perdono la casa per l'aumento del tasso dei mutui. Quindi, vediamo vediamo il nostro voto positivo su questa fiducia al Governo come un un riconoscimento del lavoro che la maggioranza ha saputo fare al Senato, pur nella consapevolezza dei limiti che permangono. Il decreto è migliore ora di quanto non fosse. Non è quello che avremmo scritto, ma è comunque migliore di quello che era. prendiamo atto. Vediamo in questo un auspicio di una futura azione di Governo più incisiva sul piano della sicurezza e più consapevole della necessità di dare risposta anche ai problemi di tante famiglie e di tanti lavoratori che in questo Paese vivono un momento per altro verso di difficoltà, per la sindrome della quarta settimana e forse anche della terza, come talvolta si dice! Anche su questi problemi bisogna dare risposte più efficaci e tempestive. *(Applausi dal

Sempre nella vita ho coltivato questa propensione a pormi di fronte ad ogni situazione, ad ogni evento, con atteggiamento dubitativo. Per questo motivo, forse, ho potuto coltivare anche poche, ma assolute certezze; una di queste riguarda il diritto per ogni essere umano alla vita, diritto ribadito da secoli in tutti i Paesi che hanno conquistato civiltà e democrazia e ribadito dalla nostra Carta costituzionale, che all'articolo 3 aggiunge: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Non dice la nostra Costituzione quale origine debbano avere i cittadini, accogliendo in tal modo le donne e gli uomini che compongono la società del nostro Paese. Da qualche tempo imperversa un dogma sicuritario. È iniziato, credo, nel novembre 2006, con la presentazione del patto per la sicurezza di Napoli. Da maggio arrivano i Patti per la sicurezza a Roma e Milano, poi Torino, Cagliari, Catania, Genova, Bari e Bologna. Il mito del patto è diventato, negli ultimi anni, un modello geometrico della politica e, allo stesso tempo, un grimaldello mediatico. È preoccupante che diritti fondamentali possano essere affidati a contratti, seppure nel diritto pubblico, che oltretutto giungono alla spicciolata. Le istituzioni hanno operato sulla base di contrattazione locale, con clausole invasive di diritti personalissimi, spesso eccezionalmente vaghe. Avvicinamento, incertezza e controllo hanno sviluppato il concetto di polizia di prossimità. Nel patto per Milano, la città «soffre della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e di nomadi». L'articolo 2 per un protocollo d'intesa che fa esplicito riferimento alla "emergenza rom" (cioè persone che sono emergenza), vuole distinguere «il fenomeno del nomadismo e quello relativo a etnie stanziali». Si dice, dunque, esplicitamente, che a Milano ci sono etnie. Nel patto per Roma si parla di «interventi risolutivi delle esigenze di contenimento delle popolazioni senza territorio»; è una definizione importante, io credo.

Adesso «popolazioni senza territorio»: una categoria di esseri umani è definita per ciò che non ha; si dà per scontato che sia priva di terra e che il territorio sia di chi vi risiede stabilmente. Conta il godimento d'immobili, divenuto etichetta identitaria: oggi qualcuno ha un'identità di possesso, appartiene a quelli "con". Gli altri, sono "quelli senza". I "senza" suscitano "esigenze di contenimento". Si usa un gergo, io credo, da guerra fredda e occorrono interventi risolutivi per l'inclusione sociale. Oggi, signor Presidente, approviamo un decreto del Governo di cui, mi permetta, molti di noi non sentivano assolutamente l'urgenza. Sentiamo piuttosto l'urgenza di provvedimenti in favore della scuola pubblica, che è sempre la cenerentola della nostra politica; interventi in favore della sanità, della sicurezza nei luoghi di lavoro (ancora oggi abbiamo avuto grandi dolori da questa mancanza di sicurezza). A mio parere, c'è l'esigenza di rafforzare, ancor più di quanto non abbiamo fatto con i nostri emendamenti, le norme che si oppongono a condotte discriminatorie che si basino su motivi etnici, religiosi, su orientamenti sessuali o su identità di genere. Soprattutto, ci opponiamo e ci opporremo sicuramente a

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nell'accezione comune, l'Italia viene ritenuta il Paese più europeista d'Europa; questo sentire, che tutti noi ormai abbiamo dentro, si traduce in comportamenti e persino in atti politici, scivola sul terreno del non rispetto delle regole che la stessa Europa ci impone.

la Costituzione della Repubblica italiana, la giurisprudenza costituzionale che si è formata, ma anche la legislazione europea; da qualche anno, inoltre, le cose non hanno più neanche un diverso valore, una diversa rilevanza.

eppure, tanti colleghi, in qualche misura, hanno cercato di modificare ciò che la normativa europea ci ha indicato a servizio di un'esigenza che tutti avvertiamo. Le parole del Ministro dell'interno, che sono risuonate in quest'Aula (un po' distratta, devo dire), assolutamente esemplari dal punto di vista dei riferimenti normativi, quando egli ci ha detto che per andare oltre bisognava cercare di modificare la direttiva europea. Tuttavia,

e che annuncia, proprio nei suoi *considerata*, come questi diritti siano assolutamente inalienabili e non modificabili perché discendono direttamente dal Trattato; abbiamo pensato di potervi porre dei vincoli attraverso una legislazione nazionale, con una palese violazione della norma costituzionale laddove avessimo acceduto a queste proposte. Eppure, signor Presidente, le posso assicurare, come unico ex relatore di questa legislatura, che tutti i tentativi di trovare un punto di convergenza con l'opposizione su un argomento come questo sono stati sperimentati, ma ogni qual volta è stato proposto un tema di condivisione se ne poneva subito uno nuovo che richiedeva necessariamente un rifiuto, perché il vincolo non era quello della buona volontà, ma era rappresentato dalla Costituzione e dalla direttiva europea.

né la libertà che ha origine dalla restrizione di ogni spazio di decisione, anche in campo politico, che abbiamo conosciuto durante i regimi totalitari.

e trovare spazi maggiori di azione. Lì deve rispondere l'Europa, Presidente, e dobbiamo rispondere noi con una cultura nuova e diversa.

Anche più recentemente, Ralf Dahrendorf ha scritto che la sicurezza per la libertà è lo *slogan* del quale dobbiamo indottrinarci se vogliamo restituire a questo Paese e alle nostre comunità quegli spazi di libertà che oggi si pretendono.

a fornire risposte europee a queste problematiche. Non possiamo nasconderci dietro un dito e non prendere atto che esiste un problema di siffatta natura. Non possiamo far finta che tutto vada bene in virtù di un egualitarismo immaginario che non c'è. Ci sono situazioni diverse che vanno affrontate con strumenti adeguati e non deve mancare, oggi, quel presidio di garanzie per la libertà che tutti noi pretendiamo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sicurezza di oggi dovrebbe essere nel cuore e nella passione politica del centro‑sinistra, dovrebbe essere il nostro modo di concepire la vita e la quotidianità. È una sicurezza ed una libertà che ci chiedono soprattutto le comunità e i cittadini meno agiati, coloro che non hanno il denaro per permettersi *bodyguard* o istituti di vigilanza privati. non ha mezzi oggi, in un sistema che dal punto di vista delle sicurezze non è sufficientemente garantito dallo Stato, è più debole dinanzi alla violenza, ed è più debole dinanzi anche alle istituzioni giudiziarie. o immaginiamo che questo Paese debba dotarsi di una maggior sicurezza e di istituzioni più forti sotto questo profilo o noi non renderemo un servizio né alle nostre libertà, né a coloro che in questo momento vivono in condizioni peggiori nel nostro Paese. Non a caso, questi temi sono meno avvertiti in centro che nelle periferie e credo che già questo dovrebbe essere uno stimolo per noi per immaginare che ci debba essere un sentiero nuovo anche del nostro pensiero, che ci debba essere un sentiero nuovo anche del nostro agire politico e che tale questione non possa essere più di destra, ma che debba essere una questione nostra, vissuta con pienezza e secondo i princìpi che io ho enunciato: la Carta costituzionale e la legislazione europea, della quale abbiamo parlato a lungo senza rispettarla in quest'Aula. Signor Presidente, voglio aggiungere, concludendo, soltanto due questioni, una di carattere generale generale e una personale. La prima di carattere generale riguarda il trasferimento delle competenze dal giudice di pace al giudice ordinario penale. Signor Presidente, io, come ex relatore, ero la persona meno adatta per sostenere la competenza penale del giudice di pace.

di pace, io sostenni allora, non per ragioni costituzionali (che peraltro sono state chiaramente superate dalla Corte costituzionale quando ha detto che non c'era un principio di irragionevolezza), per una questione di carattere sistematico ineluttabile, che quella scelta sarebbe stata sbagliata. Il legislatore italiano ha deciso che la competenza del giudice di pace dovesse essere una competenza penale, ma che non dovesse afferire la questione delle libertà personali; e quella della competenza in materia di convalida per gli extracomunitari, ed oggi per i comunitari, laddove il provvedimento al nostro esame non fosse stato modificato, sarebbe stata un'assoluta singolare originalità. Ad un giudice che abbiamo voluto specializzato per le questioni della convivenza e perché doveva dirimere il naturale dissidio che può verificarsi in una società al giorno d'oggi, veniva fatto carico dell'applicazione dell'articolo 13 della Costituzione soltanto per alcune categorie di soggetti. La sistematica impediva l'attribuzione della competenza penale in materia di libertà personale al giudice di pace, non altro; e io credo che abbiamo fatto un buon lavoro di risistemazione generale quando abbiamo restituito queste competenze al giudice ordinario penale. Concludo con una questione personale, Presidente. Ieri ho taciuto durante tutto il resto della seduta, quando si è aperta una polemica vivace su un voto incoerente rispetto a quello che avevo in qualche modo annunciato. Lei stesso è intervenuto, ma io non intendo introdurre qui alcuna questione di carattere regolamentare. Il Presidente ha deciso di affidarla alla Giunta per il Regolamento, lì verranno assunti i verbali come punto di riferimento per distinguere situazioni che io reputo assai diverse e che, comunque, dovrebbero indurre un'Aula adulta e matura a distinguere tra il diritto di parola e il diritto di voto. Premesso questo, Presidente, la cosa che ho trovato davvero singolare - lo voglio dire ai colleghi e agli amici dell'opposizione - è che, nel momento in cui io cercavo di invitare i colleghi della maggioranza ad accettare le proposte dell'opposizione, delle quali ho sempre un grandissimo rispetto, perché ho rispetto di tutte le proposte che vengono portate in quest'Aula, mentre facevo questo sforzo di comunione, di condivisione per cercare di fare in modo che alcune contrapposizioni si potessero superare su un tema che ritengo patrimonio comune di questo Paese, venivo tacciato da loro di incoerenza e di aver violato il Regolamento. Allora sì, Presidente: ammetto di essere incoerente. Sono incoerente se la coerenza è quella dei blocchi contrapposti, della mancanza di ragionamento, della mancanza di volontà di trovare un punto di vista comune. quella di mettersi la casacca o l'elmetto in testa e partire l'un contro l'altro armati, rinunciando a qualsiasi ragionamento, ebbene sì, Presidente, rispetto a quella coerenza io sono incoerente, rispetto a quel conformismo, io sono anticonformista,

intervengo per esplicitare una posizione diversa da quella espressa finora dal mio Gruppo, in ultimo dal senatore Villone che ha appena parlato - lui sì - a nome del Gruppo; una posizione diversa da quella manifestata finora dalla coalizione di centro-sinistra; una posizione molto, molto diversa da quella manifestata dalla coalizione di centro-destra. una posizione, la mia, certamente minoritaria, almeno in questo ramo del Parlamento (di ciò sono consapevole); ritengo, con molta modestia, che anche una posizione come la mia debba essere manifestata in Parlamento e debba trovare spazi negli atti dello stesso. Considero questo provvedimento, signor Presidente, onorevoli colleghi, un provvedimento sbagliato e non condivisibile. È sbagliato innanzi tutto il fatto che si sia scelta la strada del decreto-legge. Resto convinto che questioni che attengono alla sicurezza, ma anche ai diritti delle persone, di tutte le persone, alle loro individuali libertà, non possano essere affrontate con la fretta - appunto - di uno strumento come il decreto-legge e soprattutto non possano essere esaminate sotto la spinta emotiva di un tragico episodio come quello avvenuto a Roma. a Roma. Mi chiedo - lo dico senza alcuna polemica - se fosse stata altra la città, e non quella che vede il sindaco anche *leader* del maggiore partito della coalizione di maggioranza, se la scelta sarebbe stata la stessa. Mi pare che questo provvedimento non ci faccia superare il rischio che la propaganda sovrasti quello che sarebbe stato giusto fare. Se ci si fosse affidati al confronto parlamentare, dedicando ad esso il tempo necessario, non sono convinto che la proposta sarebbe stata quella di cui oggi ci stiamo occupando. E d'altronde ho appena sentito - di questo lo ringrazio - il collega Villone, del mio Gruppo, che ha chiaramente affermato che il provvedimento, se fosse stato scritto da noi, non sarebbe quello di cui ci stiamo occupando.

ma non in maniera da ritenere (almeno questa è la mia posizione) che non costituisca in molti punti una grave violazione dei diritti e delle libertà dei cittadini comunitari ed in molte parti anche della stessa direttiva comunitaria; tutto ciò senza introdurre misure effettivamente efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e degli individui.

e tali da minacciare diritti e libertà. Non condivido la soluzione trovata per i centri temporanei di accoglienza (lo voglio dire al senatore Di Lello Finuoli): la considero una scelta ipocrita, un cedimento politico, quindi, e in contrasto con il programma elettorale e con la stessa cultura politica del centro-sinistra. Questa scelta, a mio avviso, ci allontana dall'Europa, sminuisce il ruolo che l'Italia ha sempre avuto in Europa e nel mondo nella difesa dei diritti e delle libertà, ed è appunto in Europa che andava posta la questione e con l'Europa che andava trovata la soluzione, non con scelte unilaterali del nostro Paese. Tuttavia, signor Presidente, sul provvedimento al nostro esame è stata posta la questione di fiducia. Tutti sappiamo quali sono i rapporti di forza in questo ramo del Parlamento, che non consentono né voti in dissenso, né perfino la stessa scelta di non partecipare al voto, perché l'una o l'altra farebbero ricadere sulle spalle di chi dovesse assumere tale comportamento le sorti

facendo violenza a me stesso, alla mia coscienza, al mio convincimento politico e dico che questo, tra tutti quelli che ho finora espresso in Parlamento, è un voto di cui non vado fiero.

quasi la commozione, per vedere così maltrattata una cosa che considero ancora un po' una mia creatura. Lo ricorderanno anche alcuni colleghi che sono in questo Senato e che erano presenti quel 28 aprile 2004, quando, dopo un dibattito a dir poco vivace in Parlamento europeo, riuscimmo a far passare questa direttiva. Peccato che l'applicazione che ne fa il Governo sia nello stesso tempo miope e strabica.

Peccato davvero, perché la direttiva contiene indirizzi ben più completi e complessi che portano al comma 5 dell'articolo 20, quindi all'espulsione, attraverso un percorso che giustifica tale misura e in un certo senso ne crea le basi filosofiche attraverso importanti innovazioni, per esempio, sul terreno dell'acquisizione della cittadinanza europea, partendo dal principio base della libera circolazione e passando dal necessario strumento del permesso di soggiorno, che da temporaneo può diventare anche permanente.

l'ambizione che essa contiene è documentata dal fatto che ne aggiorna e ne sostituisce ben nove precedenti, oltre ad un regolamento; quindi, nella sostanza, rappresenta un testo unico destinato a durare e ad essere riconosciuto - come è riconosciuto - da tutti i Paesi membri:

Non hanno trovato, per esempio, la dovuta considerazione passi avanti storici come l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente per il cittadino comunitario e i suoi familiari dopo solo cinque anni di residenza regolare e continuativa, con un trattamento pressoché identico a quello che hanno i cittadini nazionali del Paese ospitante. Vi sono forme di tutela molto sottili e complete per i coniugi, per i figli, per il nucleo familiare; coniugi e figli anche di Paesi terzi, che con la condizione di convivere con il cittadino comunitario acquisiscono gli stessi diritti. Vi fu uno scontro furibondo sul tema della famiglia, su cosa fosse in realtà questa famiglia da tutelare e da includere in tali diritti e ci fu la solita differenziazione fra destra e sinistra. Ne emerse che, accanto alla famiglia tradizionale, anche i *partner* non sposati nei Paesi in cui la legislazione nazionale riconosce i diritti prevalenti al matrimonio, possono godere di tali prerogative. E dove non esiste tale riconoscimento, si applica l'articolo 3 della direttiva, se è a carico del cittadino comunitario. Sono grandi innovazioni; ve ne sono anche altre - purtroppo, il tempo che mi è concesso è molto ridotto che potrebbero illustrare e meglio motivare il ricorso alla direttiva, ma nel suo complesso. Mi rendo conto che al Governo serviva soltanto un riferimento per l'allontanamento, ma, così presentato e considerato, diventa esclusivamente un provvedimento di pubblica sicurezza. La direttiva guardava molto più lontano; non guardava alla pubblica sicurezza, ma alla condizione dell'uomo, del cittadino inserito in un sistema europeo.

signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, è apparso quanto mai evidente, sia dal circo mediatico dei giorni scorsi che da gran parte degli interventi che si sono alternati in quest'Aula, durante l'esame del decreto-legge sulla sicurezza, n. 1872, quanto l'Italia sia oggi cambiata, soffocata da un'emergenza criminale che c'era già e - mi sia consentito dirlo da cittadino del Nord - prima ancora dei fatti di Roma e prima ancora dell'omicidio della signora Giovanna Reggiani ad opera di un cittadino rumeno. è stato cieco il Governo, come gran parte della sinistra, a non riconoscere per tempo che la questione sicurezza aveva assunto i caratteri di una vera e propria emergenza nazionale. Nella mutata caratteristica dell'immigrazione in cui l'attuale onda di piena è stata caratterizzata dall'invasione dei Paesi europei centro-orientali, appartenenti all'Unione Europea, in nome di malintesi solidarismi e fin troppo benintesi interessi economici, si sono irragionevolmente importate non solo persone perbene, in cerca di lavoro, di prospettive di miglioramento della loro esistenza e talvolta di una Patria, ma anche carrettate di malfattori poveri e delinquenti di professione, che hanno lasciato il loro Paese perché più severo del nostro nell'applicazione delle pene e dunque destinati a cercare nella malavita la fonte della loro sussistenza. Persino il Ministro dell'interno rumeno si accanisce contro Prodi, Amato e Veltroni. Dalle pagine di un importante quotidiano, afferma fiero che nella sua Nazione nel 2007 gli stessi reati che sono incrementati in Italia risultano diminuiti del 26 e dunque la colpa di tutto ciò risiede nell'eccessivo lassismo di questo Governo e delle leggi italiane, che attraverso un inaccettabile permissivismo attraggono la proliferazione di baraccopoli e campi rom che diventano il principale ricettacolo della delinquenza. Cosa risponde al Ministro la sinistra radicale? Ancora una volta fa piegare la testa al Paese in nome del buonismo solo per difendere la delinquenza. Abbiamo sentito in quest'Aula da parte di un ex autorevole magistrato profonde riflessioni sul concetto di libertà personale che sarebbe stata violata se fossero stati approvati emendamenti dell'opposizione. Ma dove sta la coerenza e la rigorosità dei comportamenti? Forse la difesa e la tutela della libertà personale vanno usate ad intermittenza? C'è una dignità più degna da tutelare se appartiene ai rom anziché ai cittadini italiani arrestati e messi nelle patrie galere nella non dimenticata vicenda di Tangentopoli? È mancato, nella gestione di questo delicato quanto difficile passaggio dell'immigrazione, l'elemento del buon senso, virtù sempre più necessaria e sempre meno presente, che avrebbe dovuto consigliare la predisposizione di leggi meno perforabili, tribunali più solleciti, giudici meno disposti a sacrificare Abele per salvaguardare Caino e carceri meno facilmente transitabili. Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno dimostrato invece come per effetto di un fin troppo superficiale buonismo siano esplosi, affermandosi, falsi miti. Dalla spettacolarizzazione di tragedie che hanno visto protagonisti alcuni immigrati sono stati creati personaggi paradossali, carichi non di un'umanità desiderosa di integrarsi, quanto piuttosto di ideali sbagliati. L'UDC nutriva molte speranze nella definizione di un disegno di legge che, seppur tardivo, si fosse occupato con serietà e rigore di espulsioni e sicurezza. Senza la sicurezza, infatti, la società regredisce e si riempie di istinti negativi al limite del razzismo, si colora di paura, si trasforma in una giungla dove l'uomo è *homini lupus*, e le tigri sono tigri per tutti. Invece siamo qui, di fronte ad una sorta di decreto-fantasma che ha prima mostrato la faccia feroce e ha poi assunto quella remissiva: una sorta di maschera pirandelliana, indossata - verrebbe da dire - quasi ironicamente per rispondere ad un antico tabù della sinistra, più attenta alle ragioni e alle miserie di chi delinque che alle ragioni e ai diritti delle vittime. Anche il voto di fiducia posto dal Governo su questo provvedimento non rappresenta la risposta al sedicente ostruzionismo dell'opposizione, ma più onestamente la cura ai suoi mal di pancia. Tradotto, è il prezzo della resa pagato in contanti dalla maggioranza e soprattutto dalla componente moderata alla sinistra estrema per garantire la sopravvivenza sempre più incerta di questo Governo. La decretazione d'urgenza che venne posta alla base del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, non fece assumere all'UDC una condizione di pregiudiziale contrarietà, perché, all'insegna del "meglio tardi che mai", vedevamo di buon occhio il fatto che finalmente, anche dalle parti del Governo, ci si fosse accorti della necessità di intervenire a sostegno del diritto alla sicurezza, non con panni caldi, ma con provvedimenti certi. Purtroppo, con il passare dei giorni ci si è resi sempre più conto della farraginosità di un provvedimento risultato fasullo, stante l'incapacità di dare risposte immediate ed urgenti. Abbiamo più volte sollecitato il Governo e il ministro Amato, fuori e dentro quest'Aula (visto che di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno), a spiegarci perché nel decreto privo di copertura finanziaria sia stato confusamente previsto un numero oscuro di comunitari da allontanare. Sa bene, il Ministro, che non possiamo prendere per buona la motivazione secondo cui le disposizioni previste troveranno copertura negli ordinari stanziamenti previsti per le espulsioni degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

È paradossale che in questo decreto non si siano volute accogliere proposte presentate in maniera unitaria dalle forze di opposizione, che, seppure con le dovute garanzie, davano maggiori certezze e rigore all'immediato allontanamento dal territorio nazionale, in presenza di decisioni giudiziali ovvero motivi imperativi di pubblica sicurezza, verificati attraverso opportune procedure da parte di organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza dei cittadini. Sfugge alla nostra comprensione la ragione del rifiuto che avete opposto all'introduzione di norme severe nei confronti di cittadini espulsi da altri Paesi e che arrivano in Italia. Non basta appellarsi alla direttiva. Questo Governo non può continuare a mandare messaggi contraddittori al Paese. Non può continuare ad avere sulla questione della sicurezza lo stesso comportamento che ha tenuto per la questione droga, per cui il ministro della salute Livia Turco il giorno prima ha disposto l'invio dei NAS nelle scuole per controllare se i ragazzi facevano uso di droga ed il giorno dopo, con una logicità che sa solo Dio, ha elevato la soglia di cannabis consentita ad uso personale. Se sulla sicurezza il Governo, la sua maggioranza e questo Parlamento vogliono fare sul serio, allora devono dimostrarlo. Il ministro Amato deve dire chiaramente - e non lo ha fatto - quali e quante risorse vorrà predisporre per uomini e mezzi al fine di garantire l'efficacia del provvedimento. Il ministro Amato ed il Governo devono - e non lo hanno fatto - rispondere con i numeri: 1.300 euro al mese sono lo stipendio di un agente di sicurezza, sono la misura di una cifra entro la quale chi è preposto a garantire ogni giorno la sicurezza dei cittadini deve non solo vivere e mantenere la famiglia, ma addirittura deve quotidianamente giocarsi la vita! Sulla questione della sicurezza l'UDC non intende buttarla in rissa, in nome di quello che è definito il solito viziaccio italiano, ma chiede con forza alla maggioranza, a quella parte moderata qui rappresentata, di uscire dall'equivoco, di non piegarsi ai ricatti di Rifondazione Comunista e soci e della sinistra estrema che, sin dal giorno successivo all'approvazione del cosiddetto decreto sicurezza nel Consiglio dei ministri, lo hanno definito una sorta di attentato ai diritti costituzionali e, annunciando opposizioni a quelle che nelle loro fantasie sono apparse come deportazioni di massa, hanno introdotto emendamenti e condizionamenti che hanno confinato il provvedimento nella poco lusinghiera politica degli annunci.

che avesse tenuto bene a mente l'imprescindibilità dei termini legalità, sicurezza ed integrazione; invece, siamo qui a segnalare - quasi a gridare - non con rassegnazione, ma con preoccupazione la non adeguatezza ed inutilità del provvedimento che questo Parlamento si appresta ad approvare. La sinistra estrema non ha perso occasione nemmeno in questo provvedimento per incassare un punto a suo favore, mettendo nell'angolo la componente teodem e pretendendo di inserire norme che con la sicurezza hanno poco a che spartire. Che ci azzecca - per dirla con Di Pietro - nel decreto sulle espulsioni l'introduzione del reato con relativa pena per l'estensione del concetto di discriminazioni di genere? In questo provvedimento non emerge un segno netto nella direzione della legalità e della lotta vera alla criminalità.

«Lo si è fatto per che cosa?». Oggettivamente, non si capisce. Quali poteri straordinari oggi andiamo ad attribuire agli organi di polizia se un'emergenza esiste? Noi diciamo che viviamo un momento straordinario

Si va ad individuare un ordine di reati gravissimi:

Sappiamo che i provvedimenti dell'ordine magistratuale vanno indubbiamente portati a conoscenza dell'interessato, cioè notificati:

va notificato il provvedimento di un giudice che inevitabilmente le troverà irreperibili: per raggiungere quale obiettivo? Vanificare tutto quello che si voleva

aveva posto nel dialogo una delle condizioni per approvare il provvedimento. Esce anche sconfitto l'appello del Presidente della Repubblica, che aveva invitato i due blocchi presenti qui in Parlamento a dialogare, al fine di costruire un testo condiviso.

avevamo posto pochissime questioni e raggiunto anche uno schema di accordo in Commissione; chi l'ha rinnegato non è stato certamente il centro-destra. Avevamo posto poche questioni, come quella dell'obbligatorietà dell'iscrizione una volta trascorsi i dieci giorni dai tre mesi previsti per la libera circolazione del Paese.

Ebbene, non vi è stato niente da fare: la parte moderata della coalizione ha dovuto accettare, ancora una volta, il *diktat* di Rifondazione Comunista.

questo sia l'ultimo provvedimento e si apra, sin dalle prossime riforme elettorali ed eventualmente costituzionali, un dialogo nel Paese che ci porti ad uscire dal pantano in cui siamo caduti. Ma oggi i veri sconfitti sono obiettivamente i cittadini italiani che hanno posto attorno a questo decreto tante speranze affinché non si ripropongano più i gravi fatti avvenuti a Roma. Viviamo una emergenza legata alla vicenda dei rom. Non dobbiamo negarlo. Non si tratta di una questione razzista. Perché non abbiamo adottato la moratoria? Perché il Governo non ha fatto come la Germania, l'Austria, la Francia e la Spagna? Sono finiti in Italia 200.000 rom

grandemente diminuita. Questo è il vero problema di cui bisognava tenere conto. Esce sconfitto da questo dibattito anche il nostro vice presidente

del *welfare*, non potevate ingoiare anche quello di un provvedimento sulla sicurezza che fosse migliorativo rispetto alle attuali condizioni, che garantisse veramente una politica rigida in ordine agli allontanamenti dal nostro Paese.

Se voi lasciavate votare liberamente il Parlamento, sicuramente su una serie di emendamenti migliorativi potevano esserci delle maggioranze trasversali che avrebbero perfezionato il provvedimento. Invece, siete voluti andare fino in fondo nella forzatura della mano. Avete introdotto in questo provvedimento di legge delle

dovranno essere allontanati vengano tenuti nelle sale delle questure o mantenuti vicino ad esse, oppure domani con provvedimenti vadano direttamente agli arresti domiciliari.